la più bella delle figlie di Priamo, re di Troia, e di Ecuba, Cassandra, non era un uccello del malaugurio, come ritengono erroneamente alcuni che usano a sproposito i fatti e i personaggi della mitologia, bensì una profetessa inascoltata, cioè una persona capace di prevedere chiaramente la verità, ma condannata a non essere creduta. Se Priamo le avesse creduto quando sosteneva che il cavallo di legno lasciato dagli Achei sulla spiaggia era pieno di soldati nemici, sarebbe stata raccontata un'altra storia. Per quanto mi riguarda, non sono una Cassandra per vocazione: sono soltanto molto preoccupato, non solo da oggi. dal 2002 - che mettiamo in guardia sui rischi inerenti ad un mercato finanziario privo di regole certe e di trasparenza. La prima mozione da me presentata è infatti datata 27 febbraio 2002; già in essa puntavo il dito sulle bolle finanziarie e i sui rischi che comporta un liberismo sfrenato. Tutti ricordiamo le crisi bancarie del 1997 in Asia, quelle in Russia, quella dell'America Latina e, nello specifico, il crollo della *new economy* negli Stati Uniti, la gigantesca crisi bancaria giapponese del 2002 e la bancarotta dell'Argentina. I nostri appelli e quelli di molti autorevoli esperti del settore, come quello dell'economista americano Lyndon LaRouche e dei suoi seguaci, come allora in Italia Paolo Raimondi, sono purtroppo rimasti inascoltati. E anche adesso chiedo al Sottosegretario di dare un po' di attenzione al dibattito. Il risultato è che oggi ci troviamo dinanzi ad una crisi che rischia di diventare peggiore di

Ribadisco quanto detto prima: se qualcuno avesse ascoltato i nostri appelli negli anni passati, avremmo potuto evitare questo disastroso crollo economico-finanziario. Ricordiamo tutti che la grande crisi del 1929 portò la comunità internazionale a stringere gli accordi di Bretton Woods al fine di darsi regole precise per i mercati valutari e finanziari; inoltre, agli Stati fu chiesto di sorvegliare e regolamentare il mercato. Perché, allora, il sistema è andato in crisi? Per il credo assoluto in un liberismo totale dei mercati, soprattutto sulla scia del liberismo americano, a partire dagli anni Settanta,

essere ridotto al minimo. Ciò che ha causato la crisi odierna è stata dunque la mancanza di un controllo rigoroso e l'assenza di trasparenza nei bilanci delle società finanziarie e degli istituti di credito. L'economia mondiale, che in passato si basava sul lavoro effettivo, sugli investimenti in infrastrutture, su prodotti e servizi reali, dunque su una ricchezza concreta, si è trasformata sempre più in un'economia del debito, basata sulle speculazioni finanziarie e sulla crescita dei valori fittizi. Si è fatto abuso dei contratti derivati; parlo di abuso perché lo strumento è nato per tutelare l'agricoltura, ed era utile in tal senso, ma con il tempo è diventato un mostro per speculazioni ad altissimo rischio. In aggiunta a ciò, vi è stata - lo ribadisco - la totale assenza di controlli sui grandi istituti finanziari, ma anche sulle imprese. I crolli dei giganti produttivi americani (ricordiamo Enron Enron e WorldCom) manifestarono i primi sintomi di questa malattia, ma anche l'Italia, pur sotto la supervisione sui mercati svolta dalla Banca d'Italia, non è stata così virtuosa come si vuol far credere.

e di una battuta si trattava - che la nostra fortuna era quella di non saper parlare inglese. Capisco l'ironia e ciò a cui si riferiva il Ministro, ossia il fatto che nel nostro sistema non vi è stato un abuso di strumenti cosiddetti sofisticati come nell'economia anglosassone; onorevole Presidente, colleghi, non nascondiamoci dietro un dito: anche in Italia, purtroppo, il sistema finanziario ha fatto uso di strumenti speculativi, scaricando spesso sulle spalle degli investitori le perdite causate da un sistema divenuto marcio. Ricordo, in tal senso, un'analisi

Ciò che ha determinato la crisi che oggi ci troviamo a dover fronteggiare, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, sono stati i mutui *subprime*, cioè quei mutui concessi a chiunque, anche a chi non ha la capacità di onorare il debito. Con lo scopo di attirare clienti non avevano le risorse per soddisfare i termini dei contratti l'industria del credito *subprime* ha messo in atto pratiche predatorie, e le conseguenze le abbiamo viste. Anziché assumersi il rischio connesso a questo tipo di credito (normalmente una banca locale presta il denaro, si fida delle persone o controlla i propri clienti e loro possibilità di pagamento), gli istituti finanziari hanno impacchettato queste posizioni creditorie con strumenti finanziari sofisticati vendendoli in giro per il mondo. Così facendo si è perso il legame diretto di responsabilità tra chi aveva aperto il mutuo e la banca che lo aveva concesso. Questi titoli dall'incerta liquidità, definiti "tossici", sono finiti nei nostri fondi pensione, nei fondi d'investimento e nella pancia delle banche. occorre porre le basi affinché in futuro non riaccada ciò che sta avvenendo, affinché non si cada più nella trappola dell'emergenzialità. Siamo in ritardo, ma oggi più che mai è necessario riorganizzare il sistema creditizio e finanziario, e questa è la richiesta comune che trapela da tutte le mozioni presentate. Personalmente, chiedo al Governo di salvare almeno l'essenziale di questo comune appello ad un riassetto internazionale del sistema bancario, finanziario e del credito. creato dalla speculazione, però, non può essere colmato con i soldi dei contribuenti, né soltanto con misure d'urgenza. Occorre piuttosto puntare alla salvaguardia dei piccoli risparmiatori, non limitandosi ai loro depositi, ma anche tutelando i loro investimenti nei fondi pensione e nei fondi d'investimento non speculativi, ovviamente fino ad un certo limite, lasciando che il mercato ripulisca, anche in modo drammatico, il sistema finanziario dai cosiddetti strumenti tossici. Non condividiamo, dunque, quanto hanno intrapreso le autorità americane, le quali hanno utilizzato i fondi dello Stato per coprire non i bisogni delle famiglie, ma le perdite provocate dai titoli ipotecari MBS (*Mortgage Backed Securities*) e dagli e dagli strumenti derivati, che, utilizzando artificiose leve finanziarie, hanno moltiplicato i valori speculativi oltre l'immaginabile. Per fare un esempio, basti pensare che lo scopo dichiarato del salvataggio della il colosso assicurativo americano numero uno nel mondo, e di altri istituti è stato quello di garantire la copertura dei titoli derivati legati alla speculazione nel settore dei mutui *subprime*, piuttosto che

cioè quelle che si basano sull'effettiva economia reale. I titoli tossici vanno eliminati, ma, come sostenuto recentemente dallo stesso ministro Tremonti (e su questo lo appoggiamo pienamente), respingiamo l'ipotesi che lo Stato, con i soldi dei contribuenti, si faccia carico di queste perdite. In parole povere, lasciamoli fallire. È stato questo, tra l'altro, il metodo impiegato nella ricostruzione postbellica in Europa e dal *New Deal* attuato dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt durante la Grande Depressione, che permise il superamento della crisi e la ricostruzione dell'economia sia americana che europea.

e da altri senatori, puntano a sollecitare un impegno da parte del Governo italiano ad agire in sede internazionale per promuovere una nuova riorganizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale, cooperando con le principali potenze mondiali e con quelle emergenti al fine di stabilire un nuovo sistema. Il modello che proponiamo si basa su quello adottato per superare la grande crisi del 1929, ovvero il modello di Bretton Woods, come tra l'altro propongono il grande economista americano Lyndon LaRouche e molti studiosi come Andrew Spannaus. Per uscire da questa crisi e far ripartire la ruota dell'economia dobbiamo innanzitutto ripristinare la fiducia nei mercati finanziari, e questa fiducia si ripristina con regole certe e trasparenza (condizioni imprescindibili per dare credibilità al sistema) e con un'amministrazione controllata del sistema bancario, diversificando e separando i debiti speculativi da quelli di investimento. I debiti speculativi rappresentano purtroppo la stragrande maggioranza dei valori che gravano sui bilanci delle principali banche commerciali e di investimento, e, come giustamente sottolineato dal ministro Tremonti, persino sui bilanci di certi enti locali italiani. La fiducia non si ottiene se questi debiti speculativi vengono salvati con i soldi dei contribuenti. La fiducia si ottiene se c'è giustizia, se pagano coloro che li hanno messi in circolazione. Il salvataggio, dunque, deve Il salvataggio, dunque, deve concentrarsi sulla garanzia degli investimenti dei piccoli risparmiatori. Questa garanzia non si deve limitare ai depositi bancari, ma deve comprendere - fino ad un certo limite - anche i fondi pensione e i fondi comuni d'investimento non speculativi. Prendiamo nuovamente l'esempio americano: piuttosto che comprare i titoli tossici dei mutui *sub**prime*, il Governo americano avrebbe potuto utilizzare i propri fondi per comprare gli immobili stessi, proteggendo così i piccoli risparmiatori e le famiglie indebitate. Anche l'Italia deve differenziare: non si può salvare con i soldi pubblici il marcio, con il rischio di non avere più fondi per aiutare i nostri risparmiatori, le nostre famiglie, le nostre imprese. Il sistema riconquista credibilità se al bene comune, al *general welfare*, viene data precedenza assoluta rispetto agli obblighi creati per foraggiare la bolla speculativa e per ottenere in breve tempo facili e cospicui guadagni. la fiducia si ottiene se si garantisce più stabilità alla produzione e al commercio internazionale. Sono dunque necessari cambi valutari cambi valutari più stabili e non lasciati al mercato, ma decisi con accordi tra le nazioni evitando le oscillazioni speculative dei mercati. Apro una parentesi. Un imprenditore italiano che vende i suoi prodotti in America non dovrebbe essere esposto, come purtroppo è stato in questi anni, alle fluttuazioni del dollaro, pagando così i debiti contratti dagli Stati Uniti per finanziare le loro guerre. Con l'immissione di liquidità gli americani mirano ad una ulteriore svalutazione del dollaro (anche in questi giorni), facendo così pagare nuovamente all'economia europea in generale e agli esportatori in particolare il loro debito. Per dare stabilità è infine necessario aumentare i controlli sui trasferimenti di capitali a fini speculativi, ovvero ripristinare il *capital* *control*, privilegiando gli investimenti a lungo termine nell'economia produttiva. produttiva. Condividiamo, a tal fine, quanto detto dal ministro Tremonti, ossia privilegiare, nel sistema creditizio, con un basso tasso di interesse e a lungo termine, gli investimenti in infrastrutture, industria ed alta tecnologia, piuttosto che incoraggiare la ricerca del profitto facile a scapito dell'attività produttiva. La fiducia si ottiene se il sistema creditizio diviene effettivo e non puramente monetario. Questa è stata, tra l'altro, l'idea ispiratrice del modello di Bretton Woods. Dalla crisi usciamo se si trova un accordo non solo con le principali potenze mondiali del G8, ma anche con le nuove potenze economiche

altri 40-50 anni. Per questo nella nostra mozione chiediamo al Governo italiano di esercitare pressioni sulla comunità internazionale e di farsi nobile promotore affinché si pongano le basi per una cooperazione internazionale capace di realizzare gli obiettivi proposti. Concludo. Riteniamo non sia sufficiente curare soltanto i sintomi della malattia, ma ciò che l'ha causata (per questo ho cercato di motivarla), ossia il sistema finanziario internazionale nel suo complesso. Chiediamo di tenere sott'occhio l'obiettivo di investire i mezzi pubblici, non per salvare i debiti speculativi, ma per proteggere i piccoli risparmiatori, le nostre imprese, le famiglie e i posti di lavoro. Chiediamo, insomma, che non sia il contribuente, la famiglia italiana a pagare due volte: una volta con la perdita dei propri risparmi o la loro svalutazione, un'altra volta con le tasse e il debito prodotto da speculazioni finanziarie.

e di giorno in giorno le notizie, anche quelle di ieri e di oggi, acuiscono le preoccupazioni. Non a caso la si paragona con la grande crisi del 1929, che causò un impoverimento globale durato diversi anni, con costi sociali e conseguenze di portata storica rilevantissimi. Di quella crisi allora le autorità non colsero per molto tempo la portata; oggi, invece, tutti i Governi e le varie autorità preposte sono pienamente consapevoli di trovarsi in un momento di gravissima crisi: semmai, non ne sa valutare fino in fondo la profondità e non si sa nemmeno se e quando entreranno in crisi altri pezzi del sistema finanziario come, ad esempio, le carte di credito e, più in generale, gli strumenti del credito al consumo. La caratteristica inquietante e drammatica del momento che viviamo è proprio l'incertezza assoluta sulle sue dimensioni quantitative: nessuno sa fin dove effettivamente si estenda e fin dove possa spingere i suoi esiti dirompenti. Alla base di questa situazione vi sono grandi responsabilità, in ragione delle scelte di politica economica e monetaria compiute innanzitutto dal Governo degli Stati Uniti e dalla Federal Reserve, che hanno mantenuto i tassi di interesse artificialmente troppo bassi per lungo tempo, al fine di sostenere l'economia e spingere i consumi, e a ciò non a caso aggiungendo la diminuzione dei controlli sul funzionamento dei mercati finanziari e l'introduzione di nuove regole, come quelle che hanno abbattuto il muro che opportunamente divideva le banche d'affari dalle banche di credito ordinario. L'eccesso di liquidità che così si è indotto si è indirizzato alla ricerca di guadagni di breve periodo, dando luogo ad una serie continuativa di bolle speculative in tanti settori. Così l'innovazione finanziaria è stata usata spregiudicatamente per distribuire gran parte del rischio sulle masse degli investitori ignari, producendo così, insieme ai danni diretti su quei milioni di persone, la più grande crisi di fiducia degli ultimi decenni e un fortissimo aumento del rischio per l'intera economia mondiale. Questo è, in sintesi, quanto è avvenuto e quanto sta avvenendo. Ma come si può rimediare e porre un argine ai danni che sono stati provocati? Molti Governi, quello americano soprattutto, in questi mesi hanno operato massicci interventi di breve di breve periodo per evitare che la crisi peggiorasse e si diffondesse sempre più il panico, ma c'è e ci sarà soprattutto bisogno di interventi con una visione di lungo periodo. Un mondo globalizzato ha bisogno di istituzioni internazionali forti, sia per gli aspetti più legati alla politica, sia per quelli propri dell'economia, perché mercati globali hanno bisogno di regole globali che i singoli Paesi potranno poi adattare alle varie specificità di ciascuno, restando tuttavia legati a una base comune. Se siamo precipitati in una crisi di cui ancora non conosciamo gli aspetti quantitativi né la durata è proprio perché negli ultimi dieci anni sono state allentate le regole e i controlli. Ciò a dispetto del fatto che in molti Paesi le autorità di controllo si sono moltiplicate, ma proprio queste moltiplicazioni hanno reso i controlli meno efficaci, isolando e dividendo i vari mercati; sono controlli che hanno soprattutto mantenuto un carattere nazionale, mentre i mercati finanziari sono diventati mondiali. È quindi interesse di tutti operare per regole e sorveglianze più severe a livello internazionale. Non sarà una battaglia facile: vediamo quanta fatica facciano le dichiarazioni d'intenti a tradursi in proposte e norme concrete. Per questo nella nostra mozione noi chiediamo che il Governo si adoperi per un nuovo disegno di regolazione dei mercati finanziari, per una riforma delle principali istituzioni di livello internazionale, per nuovi strumenti di governo dell'economia e delle società globali, a partire dalla proposta di istituire in sede ONU un nuovo Consiglio per lo sviluppo sostenibile in cui siedano permanentemente i rappresentanti delle grandi macroaree protagoniste dell'economia mondiale, e - non meno importante - di adoperarsi perché siano applicate sanzioni a carico dei paradisi fiscali, che perturbano ed inquinano i mercati. Così pure bisogna resistere alle tentazioni di chiusura e protezionismo. Questo è un aspetto di grandissima importanza perché, nell'impatto drammatico della crisi sulle economie reali, con i riflessi pesanti di recessione e aumento della disoccupazione, il rischio di risposte di tipo prettamente difensivo potrebbe imporsi, come se tutte le cause della crisi economica fossero in qualche modo riconducibili all'apertura dei mercati internazionali. E d'altra parte, se è un errore demonizzare la globalizzazione, bisogna però agire per contenerne gli eccessi e proteggere chi si trova nelle posizioni più deboli. Per questo, in coerenza con le conclusioni del recente G7 di Roma, nella mozione sollecitiamo una ricapitalizzazione su scala europea del settore bancario, una nuova una nuova regolamentazione dei mercati finanziari e un ruolo più incisivo della Banca centrale europea, un coordinamento su scala europea della gestione dell'emissione dei titoli del debito pubblico dei Paesi dell'Eurogruppo, nonché l'emissione di *eurobond* sul merito di credito dell'Unione per piani straordinari di investimenti infrastrutturali. Queste azioni si debbono aggiungere alle decisioni che la maggior parte dei Governi ha già intrapreso per immettere risorse pubbliche per la stabilizzazione del credito e del sistema economico. La mozione che presentiamo esprime però anche una forte richiesta per l'adozione di iniziative che siano di sostegno per l'economia reale per contrastare una crisi davvero pensantissima per i lavoratori, le imprese e le famiglie del nostro Paese. La nostra mozione, tra l'altro, richiama la necessità di adottare, concordando con i partner europei le modificazioni al Patto di stabilità e crescita che sono necessarie, una serie di iniziative volte a garantire l'accesso al credito (in particolare per le piccole e medie imprese), a salvaguardare i piccoli risparmiatori, a sviluppare una nuova manovra finanziaria

di «ritorno alla produzione», intendendo con questo un ritorno di importanza della produzione sia agricola che industriale. Il «ritorno alla produzione» non sarà privo di conseguenze politiche anche nei Paesi occidentali, in primo luogo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e negli altri Paesi ad alto livello di sviluppo, oltre che nel rapporto con le economie dei Paesi emergenti. Cambieranno gerarchie planetarie, modelli di consumo, stili di vita. In Europa questo sforzo di ritorno all'industria, un'industria molto più attenta ai problemi dell'energia e dell'inquinamento e alla domanda in continuo aumento nei settori della salute e delle scienze della vita, sarà diversa da Paese a Paese, perché estremamente diverso è già oggi il ruolo dell'industria dei differenti Paesi europei. Dunque, si pone anche per l'Italia, in questo quadro, in questo scenario, in questa proiezione, il tema di come rispondere alle criticità del momento e impostare quelle riforme di sistema che siano utili a farci trovare preparati quando la crisi invertirà la tendenza e le economie dei diversi Paesi riprenderanno slancio. Ci saranno opportunità e rischi che produrranno nuovi posizionamenti nel quadro dell'economia globale e che saranno anche la conseguenza di come sarà stata affrontata la fase più acuta della crisi che oggi stiamo conoscendo e attraversando. Per queste ragioni insistiamo sulla inadeguatezza delle misure finora adottate da parte del Governo e sulla necessità indifferibile di tutelare le posizioni sociali più deboli, nonché di adottare con urgenza le iniziative volte a garantire l'accesso al credito per le imprese, nel quadro di una manovra finanziaria aggiuntiva